Comunico che in data 11 novembre 2021 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP» Comunico che in data 11 novembre 2021 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze* «Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche» L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento sul disegno di legge di bilancio». Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente,

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo perviene alle seguenti conclusioni. Per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, soggiace a una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-*bis*, lettera *c)*, e 12-*quater*, lettera *a)*, della legge n. 196 del 2009. Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2021. In definitiva, si segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 202 miliardi per il 2022, dovuto a entrate finali pari a 628 miliardi e spese finali pari a 830 miliardi. Nel 2023 il saldo netto da finanziare è pari a 179 miliardi per effetto di entrate finali per 638 miliardi e spese finali pari a 818 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 116 miliardi con le entrate finali che si attestano a 645 miliardi e spese finali a 761 miliardi. Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che nel 2022, le entrate finali per la Pubblica Amministrazione sono pari a 891 miliardi, le spese finali ammontano a 996 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 105 miliardi; nel 2023 le entrate finali sono pari a 926 miliardi, le spese finali ammontano a 1.002 e l'indebitamento si attesta su 76 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 934 miliardi, le spese finali ammontano a 1.001 e l'indebitamento si attesta su 66 miliardi. Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2021, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2022. Si propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, va ricordato che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si segnalano le seguenti disposizioni: l'articolo 58, che introduce la possibilità di procedere anche in via telematica all'esame congiunto della situazione relativa alla tutela dei lavoratori nel caso della comunicazione di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro; l'articolo 59, che interviene sull'individuazione della sede INPS competente a concedere le integrazioni salariali ordinarie; - l'articolo 64, che introduce la possibilità dell'esame anche in via telematica della situazione aziendale nel caso di consultazione sindacale a seguito di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale; - l'articolo 90, comma 2, che prevede il differimento al 31 dicembre 2022 del termine per l'utilizzo dell'App-immuni e della piattaforma relativa; - l'articolo 93, comma 3, che affida alle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie compiti di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software.* Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari. Inoltre, non si rinvengono nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale. Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, esaminato il disegno di legge di bilancio per il 2022, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, preso atto della posizione del Governo, comunico che il disegno di legge di bilancio appare nel complesso in linea con le prescrizioni della legge 31 dicembre 2009 n. 196, di contabilità e finanza pubblica, fatta eccezione per le disposizioni segnalate nel predetto

pluriennale per il triennio 2022-2024) alla 5a Commissione in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni in sede consultiva dovranno comunicare i propri rapporti alla 5a Commissione entro martedì 23 novembre. Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi o ad integrare i propri ordini del giorno. La Conferenza dei Capigruppo ha rimodulato il calendario della settimana corrente e approvato il calendario dei lavori fino al 25 novembre. Nella seduta di oggi il Presidente renderà le comunicazioni ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4,

libertà sindacale del personale militare, approvato dalla Camera dei deputati; decreto-legge capienze; decreto-legge in materia di giustizia e proroghe, approvato dalla Camera dei deputati. La settimana prossima sarà riservata ai lavori delle Commissioni, che dovranno comunicare i propri rapporti sul disegno di legge di bilancio alla 5a Commissione permanente entro martedì 23 novembre. Nella mattinata di giovedì 25 novembre l'Aula del Senato sarà impegnata per un'iniziativa celebrativa della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'Assemblea potrà essere convocata giovedì 25, alle ore 16, per la discussione dei disegni di legge per il contrasto delle molestie sui luoghi di lavoro, ove conclusi dalle Commissioni. I Capigruppo hanno stabilito che, a partire dalla prossima chiama per la fiducia al Governo, verranno ripristinate le modalità di votazione con appello nominale vigenti prima dell'emergenza da Covid-19, anche ad evitare incresciosi episodi come quello che la settimana scorsa ha riguardato il senatore Bagnai. Pertanto, ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario esprimerà ad alta voce il proprio voto passando sotto il banco della Presidenza.

il MoVimento 5 Stelle ritiene che la trasparenza sia alla base della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; la trasparenza deve perciò contraddistinguere l'operato della classe politica per alimentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. C'è una vicenda che da giorni è oggetto di attenzione da parte dei *media* e che ha contorni opachi e certamente poco trasparenti; una vicenda che chiama in causa esponenti politici di rilievo e si inserisce nell'ambito dell'inchiesta sulla fondazione Open. Negli atti di questa inchiesta si prospetta infatti un vero e proprio dossieraggio ai danni del MoVimento 5 Stelle e di suoi esponenti di rilievo. In una *e-mail* inviata nel 2017 dal giornalista Rondolino al senatore Renzi, di cui allora era consulente, si legge infatti: «Caro Matteo, eccoti un primo appunto sulla struttura di propaganda antigrillina». «Sarebbe utile vederci per iniziare la Lunga Marcia». «Notizie, indiscrezioni e rivelazioni mirate a distruggere la reputazione e l'immagine pubblica di Grillo, Di Maio, Di Battista, Raggi, Casaleggio Travaglio e Scanzi». Per realizzare questo bisogna «creare una piccola, combattiva redazione» con «due giornalisti di inchiesta e un investigatore privato di provata fiducia e professionalità (a costo medio-alto)». Questa *e-mail* fu poi inoltrata dal senatore Renzi al suo collaboratore Marco Carrai. Signora Presidente, chiaramente la magistratura farà il suo corso, ma quello che stupisce me lo faccia dire - è il silenzio totale delle altre forze politiche su questo tema. Non una parola di biasimo, non una richiesta di chiarimenti, non un cenno di solidarietà nei nostri confronti, nei confronti di colleghi che siedono in quest'Aula e che sembrano essere stati oggetto di quel dossieraggio. Un silenzio che sta diventando imbarazzante. Il tema della trasparenza si collega anche ai lauti compensi come conferenziere che il senatore Renzi pare ricevere da soggetti italiani e internazionali: dimostrazione plastica del rischio che il confine tra politica e affari, tra cosa pubblica e tornaconto personale si può assottigliare fino a scomparire. Quindi, a tutti presenti e a tutte le forze politiche chiedo il massimo impegno affinché parole come disciplina, onore e trasparenza siano realmente applicate. A questo riguardo, signora Presidente, dovremmo adottare un codice di condotta per i senatori che metta al centro la trasparenza, così come è già stato fatto alla Camera, perché in questo momento storico serve un segnale chiaro al Paese. Del resto, anche l'organo del Consiglio d'Europa che si occupa di lotta alla corruzione ha sollecitato il nostro Paese ad adottare una vera e seria legge sul conflitto di interessi. Una legge sul conflitto di interessi targata MoVimento 5 Stelle è in discussione alla Camera, mentre un altro disegno di legge è stato qui depositato dal nostro collega Ferrara. Allora lavoriamoci insieme, confrontiamoci, acceleriamo e dimostriamo ai cittadini che la politica e il Parlamento hanno la forza e la volontà di rimuovere le opacità e le zone grigie di cui il nostro Paese e Il MoVimento 5 Stelle, oltre a chiedere di adottare un codice deontologico e di appoggiare la nostra proposta sul conflitto di interessi, ha anche chiesto, in Commissione di vigilanza Rai, l'audizione dell'amministratore delegato, proprio per chiarire i rapporti del nostro servizio pubblico con i soggetti imprenditoriali coinvolti in questa inchiesta. Vorrei avanzare un'altra richiesta, un'esortazione al senatore Renzi a non fare richiesta di immunità. *(Applausi)*. Del resto, era lo stesso senatore che qualche anno fa si...

Il senatore Renzi si diceva contrario all'immunità. E allora: adozione del codice deontologico, approvazione della legge sul conflitto di interessi e non ricorso all'immunità da parte del senatore Renzi. Queste sono le proposte del MoVimento 5 Stelle davvero il confronto democratico, perché senza coscienza morale il nostro Paese non ha futuro.

Noi abbiamo lasciato parlare senza interrompere, presidente Taverna. PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato tutti in silenzio. Adesso ascoltiamo quello che dice il presidente Faraone. Prego. Inviterei la presidente Taverna a non ritornare ai vecchi fasti. Ci piaceva forse di più in quel modo. Sinceramente vederla composta oggi, vederla fintamente composta oggi fa un po' ridere. Però, Presidente, quello che vorrei dire in maniera molto tranquilla e vorrei anche sottolineare è l'aspetto di chi, con l'intervento di oggi, ha chiesto solidarietà. È abbastanza ridicolo, Presidente, che il MoVimento 5 Stelle stia chiedendo alle forze politiche presenti in quest'Aula solidarietà

di destra e di sinistra, hanno subito dal MoVimento 5 Stelle quello che la senatrice Castellone sta dicendo di aver subito, cioè

Pregherei di far parlare il presidente Faraone, per cortesia. Questo modo di dissentire non fa parte della dialettica parlamentare; ognuno può dire quello che crede. Presidente, abbiamo subito, tutti noi parlamentari di tutte le forze politiche, di destra e di sinistra, la creazione di profili falsi su Facebook da parte del MoVimento 5 Stelle

stati utilizzati come manganelli nei confronti di donne e uomini perbene da una forza politica

Sinceramente, non accetto di sentir loro chiedere solidarietà per qualcosa che non è stato fatto, se non da loro, nella storia della Repubblica italiana. nella storia della Repubblica italiana. *(Applausi)*. L'unico movimento che è cresciuto con l'uso del manganello mediatico si chiama MoVimento 5 Stelle.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

Signor Presidente, intervengo dopo questa poco piacevole diatriba tra alleati di Governo che ci vede spettatori. Ad entrambe le parti avremmo qualcosa da dire, ma ci concentriamo su cose molto più importanti. Vorrei stigmatizzare quanto sta accadendo nel mio territorio, nella Provincia di Belluno, con due imprese, la ACC e

dello Stato, attraverso Fincantieri, che metta in sicurezza gli 800 posti di lavoro che oggi risultano a rischio. Ricordo

il Comune di Borgo Valbelluna, che ha un sindaco coraggioso, ma quasi logorato dal grandissimo lavoro che sta compiendo e a cui va tutta la mia solidarietà. Questo sindaco non è nemmeno della mia parte politica, è esattamente dell'altra parte, ma gli riconosco una grandissima capacità di

di tempo sia non dico doveroso, ma quanto mai gradito. Signor Presidente, dunque la ringrazio e faccio appello al ministro Giorgetti affinché chiuda questa benedetta situazione, attraverso l'intervento di Fincantieri, per quanto attiene alla ACC

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché ieri è stato pubblicato il «XII Atlante dell'infanzia a rischio in Italia», a cura di Save the Children, il primo dell'era post-Covid. Il quadro devastante che ne emerge si inserisce in una situazione di fragilità per il nostro Paese, che merita sicuramente l'attenzione di tutto il Parlamento

d'Italia. Fra pochi giorni, il 20 novembre, ricorre la Giornata mondiale dei diritti dei bambini. Ebbene, quando giusto trent'anni fa,

Ieri ho partecipato a una riunione con l'ASI di Brindisi, l'Associazione per lo sviluppo industriale della città e di tutto il territorio brindisino, e a questo proposito ringrazio anche il neopresidente Vittorio Rina del lavoro che sta svolgendo; abbiamo posto l'attenzione su alcune particolarità. Innanzitutto, è importante dire che, anche se molto spesso a proposito della Puglia sentite parlare delle problematiche che riguardano un'altra città, Taranto, anche Brindisi ha bisogno di molta attenzione.

prima di tutto rendere attrattivo il territorio, e quindi supportarlo per creare delle infrastrutture, altrimenti chi verrà ad investire in quella zona già particolare? Un'attenzione particolare deve essere data al sito SIN che deve essere bonificato, perché quelli sono i terreni messi a disposizione.

la recente apertura della questura e dei comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di finanza nella Provincia di Barletta-Andria-Trani sembra aver attenuato solo in parte il problema della criminalità in quel territorio. La BAT, tra l'altro, è confinante con Corato, l'ultimo paese della Città metropolitana di Bari, che è risultato uno dei paesi in cui si assiste al maggior numero di furti d'auto, a cui si aggiungono altri tipi di reati.

L'ultima recente notizia è quella dei sequestri lampo a scopo di estorsione, sebbene anche di poche ore, nei confronti di imprenditori. Questo dato deve fare ulteriormente riflettere su quanto su quanto l'asticella della criminalità si stia alzando. Sensibilizzo, pertanto, tutte le istituzioni competenti, i prefetti le Forze dell'ordine, a rispondere anche al grido d'allarme che è stato lanciato dal procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti, che ha consegnato alla stampa un *reportage* contenente tutte le indicazioni precise della situazione che sta investendo la BAT e il circondario del tribunale di Trani.

al fine di arrivare a una soluzione e soprattutto dare serenità a coloro che vivono in questi territori. Presidente, soltanto pochissimi giorni fa in quest'Aula abbiamo votato e convintamente approvato il prolungamento della nostra Commissione di inchiesta sui fatti del Forteto. Lo abbiamo fatto penso per motivi diversi, ma tutti quanti convinti che non si possa ulteriormente tollerare quella che è una maniera ormai sistematica di colpire i diritti dei bambini. Sabato prossimo, il 20 novembre, sarà il trentesimo anniversario della Convenzione ONU Il tema vero è che si sommano, ai danni di questi ragazzi, violenze che a volte maturano nel contesto familiare a violenze non meno gravi - a mio avviso anche più gravi - che maturano in un contesto istituzionale o para-istituzionale, come i fatti del Forteto confermano di giorno in giorno, mano a mano che il nostro approfondimento prosegue. La cosa drammatica, Presidente, che pongo alla sua attenzione è che, se il Forteto rappresenta una storia che si è conclusa - male, ma si è conclusa, perché con sedici suicidi di adolescenti e di giovani possiamo francamente dire che si è conclusa male - oggi si ripetono fatti ed eventi simili, non in maniera

questi ragazzi vengono poi affidati al genitore inizialmente accusato di violenza. Come a dire: una madre rimprovera o comunque denuncia un padre per i giochi erotici, per non parlare di violenza, con la figlia; dopodiché, dopo una lunga permanenza, confusa e pasticciata, nelle case famiglia, la bambina viene affidata al padre, ignorando le istanze che riguardano la possibile disponibilità dei nonni e tante altre cose. Sembra quasi che questi lavori non ci insegnino nulla. Io mi chiedo come sia mai possibile che il Ministero della giustizia non risponda mai alle nostre interrogazioni su questi punti e non senta mai il bisogno di fare chiarezza su situazioni che hanno un indice di drammaticità non immaginario o immaginifico, ma reale, concreto e documentato.